Presidente, vorrei pregarla di disporre la sospensione dell'esame del disegno di legge che introduce nel codice penale l'articolo 613-*bis* e il reato di tortura per consentire la presentazione in Aula di ulteriori emendamenti. La pregherei, pertanto, quando si arriverà

che tra una settimana l'ANAS inizierà i lavori della galleria di Bagnara Calabra, tagliando in due l'Autostrada del Sole. La Regione siciliana, attraverso il suo assessore, onorevole Misuraca,

intervenire presso l'ANAS affinché possa parlamentare, cosa che non ha fatto fino ad oggi, con il Governo regionale siciliano. La Sicilia non può rischiare di rimanere isolata, è già isolata

perché, peraltro, oltre ai disagi che sono stati testè esposti dal collega Strano, esiste anche un problema di correttezza nei rapporti con il Parlamento da parte del Governo. sembra che sia allo studio del Ministero un piano per sopperire ai disagi che prevede un investimento di 300 milioni di euro, il che significa investimenti duraturi.

legge n. 1678*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor rappresentante del Governo, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2006 è costruito, per la parte relativa al conto del bilancio, secondo la struttura di quest'ultimo in sede previsionale, facendo cioè riferimento alle unità previsionali di base e ai centri di responsabilità. La Corte dei conti ha tuttavia posto l'accento sulle problematiche inerenti la classificazione del bilancio, lamentando come non vi sia neanche, per l'esercizio 2006, la soddisfacente attuazione della legge 3 aprile 1997, n. 94, che mirava, attraverso l'istituzione delle unità previsionali di base, al potenziamento degli strumenti di Governo della finanza pubblica da un lato e alla misurazione qualitativa dei risultati ottenuti dall'altro. Da questo punto di vista, alla luce delle considerazioni della suprema magistratura contabile, assume un particolare rilievo l'annunciata riforma della sessione di bilancio e in particolare la riclassificazione dello stesso bilancio. L'organo di controllo auspica che la nuova classificazione non sia un mero esercizio, appunto, riclassificatorio ma uno strumento per il miglioramento dell'efficacia della spesa. L'attuale classificazione in unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativi avrebbe dato vita ad aggregazioni di spesa per lo più formali e scarsamente rappresentativi, nonché poco misurabili dal punto di vista qualitativo nell'articolazione delle politiche pubbliche. La realizzazione di un modello di riforma fondato sul principio di programmazione per obiettivi necessiterebbe, invece, dell'introduzione di un indicatore di prodotto e di impatto all'interno delle note preliminari di bilancio coerenti con le direttive generali di inizio anno. Non è possibile, dunque, con gli attuali strumenti, ancora, effettuare la prevista valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e spesa che la stessa legge 3 aprile 1997 n. 94 prevedeva, attraverso la classificazione funzionale delle funzioni obiettivo. È dunque di cruciale importanza la riclassificazione relativa al bilancio 2008 e al triennio 2008-2010, annunciata con la circolare della ragioneria generale dello Stato e discussa e confermata in audizione alle Camere dal ministro Padoa-Schioppa, che prevede, sulla base della cornice legislativa vigente, l'utilizzo di una nuova classificazione che innova profondamente la precedente struttura basata su centri di responsabilità. Il progetto di bilancio sarà organizzato in 34 grandi missioni pubbliche e in 169 programmi: la costruzione dello schema di distribuzione delle risorse da assegnare ai singoli Dicasteri di spesa parte dalle missioni e dai programmi per poi saldarsi ai centri di responsabilità.

pari a 49.983 milioni di euro. Desidero richiamare la vostra attenzione sulla circostanza che si tratta del migliore dato positivo della serie storica 1993-2006; dato assume particolare rilievo se confrontato con quello dell'anno 2005, che mostrava, invece, un saldo positivo pari a 1,5 miliardi di euro, che rappresenta, invece, il peggior dato positivo della medesima serie storica. Da rilevare, inoltre, lo scostamento, in questo caso assai significativo, tra dati di previsione definitiva che stimavano un risparmio pubblico negativo pari a -8.512 milioni di euro. Il saldo netto da finanziare, per quanto riguarda il risultato complessivo della gestione di competenza 2006, si attesta con un avanzo pari 12.949 milioni di euro (erano 21.555 e 35.210 gli analoghi dati in termini di disavanzo negli anni rispettivamente 2004 e 2005). Tale dato evidenzia un netto miglioramento rispetto all'andamento medio, anche per quanto riguarda le previsioni che, come è noto, stimavano un saldo netto da finanziare in disavanzo pari a 45.004 milioni di euro. Il dato che riguarda il ricorso al mercato finanziario, che scaturisce dal saldo tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese complessive, mostra nel 2006 un risultato che si attesta con una negatività di 150.671 milioni di euro (nel 2005 l'analogo dato era di 203.523 milioni di euro). Da notare anche in questo caso un forte scostamento tra previsioni definitive e dato consuntivo con una differenza anche qui in positivo rispetto alle prime, pari a 83.458 milioni di euro. Il netto miglioramento del ricorso al mercato è reso ancora più evidente se rapportato al saldo massimo indicato nell'ultima legge finanziaria, che prevedeva all'articolo 1, comma 1, un limite massimo di ricorso al mercato finanziario di 244.000 milioni di euro. Nel confronto con i dati gestionali, lo scostamento registrato per quanto riguarda le entrate finali tra previsioni definitive e il volume accertato è stato pari +45.666 milioni di euro, con una notevole differenza sia con le previsioni definitive (+10,5 per cento), sia con il dato del 2005 che vedeva un differenziale di +4.796 milioni di euro,

Il raffronto del dato di spesa finale (cioè spese correnti più spese in conto capitale), quale previsione definitiva confrontata con la gestione, evidenzia uno scostamento di valore di -12.288 milioni di euro, cioè il 2,5 per cento rispetto alle previsioni. Il dato assoluto delle spese finali è pari a 467.093 milioni di euro, mentre le spese complessive, maggiorate cioè dal rimborso dei prestiti, sono pari a 630.713 milioni di euro. Si sottolinea, per quanto riguarda i dati complessivi della gestione di cassa, che al netto delle regolazioni contabili il risparmio pubblico presenta un dato positivo per 4.552 milioni di euro; era 16.144 nel 2005. Il saldo netto da finanziare è pari a 25.484 milioni di euro (a fronte dei 43.836 del 2005), mentre il ricorso al mercato ammonta, in valore assoluto e sempre al netto delle regolazioni contabili, a 189.662 milioni di euro (era di 222.853 milioni di L'analisi economica delle spese finali, cioè nel dettaglio dei pagamenti, mostra, com'è noto, un aumento delle spese correnti, aumentate a 421.831 milioni di euro

rispetto al 2005), a fronte di spese in conto capitale scese a 37.972 milioni di euro, cioè meno 10,6 per cento rispetto al 2005. Nell'ambito della spesa corrente, la componente prevalente è da imputarsi alle spese di funzionamento, tra le quali prevalgono le spese per redditi da lavoro dipendente, che salgono quasi del 10 Un importante aumento sta nei trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, che crescono del 5,6 per cento. Un'ultima considerazione sul fenomeno dei residui di cassa, la cui situazione partiva all'inizio dell'anno da una differenza positiva tra residui attivi e residui passivi, e si è andata, invece, via, via modificando per effetto delle operazioni di riaccertamento, per cui al 31 dicembre 2006 vi erano residui attivi per 82.695 milioni di euro e passivi per 108.112 milioni di euro. Al riguardo occorre sottolineare il permanere, anche per l'esercizio 2006 e nonostante un decremento di un terzo rispetto al 2005, di una rilevante quota di residui attivi, sui quali sarebbe opportuna un'accurata valutazione in ordine alla loro effettiva esigibilità. Dal punto di vista del patrimonio va ricordato che l'eccedenza passiva, ossia la differenza tra le passività e le attività, è stata superiore al 4,8, con un peggioramento di circa 64 miliardi di euro. Complessivamente l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sale quindi al 4,4 per cento del PIL, ma sarebbe del 2,4 per cento del PIL al netto degli oneri per il pagamento della sentenza dell'Unione europea in materia di detraibilità dell'IVA. Il provvedimento attesta, quindi, un decisivo miglioramento dei conti pubblici intervenuto nel corso dell'anno, anche se permangono perplessità, sollevate dalla Corte dei conti sulla lettura del bilancio, in cui, ad esempio, si regista un incremento del fenomeno delle eccedenze di spesa. Le eccedenze rappresentano, com'è noto, una patologia del sistema, che riguarda, come nota il procuratore generale della Corte dei conti, tendenzialmente sempre gli stessi capitoli. A prescindere, pertanto, dai problemi sostanziali connessi all'eccesso di spesa, le cui motivazioni sono da rinvenire in decisioni assunte nel passato, si prende comunque atto, nell'ottica di un ordinato e trasparente sviluppo della gestione annuale del bilancio, dell'opportunità di una più precisa quantificazione delle effettive necessità da finanziare, relative anche alle voci di spesa per le quali il fenomeno delle eccedenze si presenta più frequentemente per importi più cospicui. Per altre e più approfondite analisi si rimanda alla lettura della nota prodotta dal Servizio di bilancio del Senato della Repubblica. e al fine di completare l'analisi sul rendiconto dopo gli interventi svolti dai colleghi nella Commissione competente, anche nell'ottica più generale che vede nel rendiconto lo strumento principe allo stato disponibile per la verifica della situazione della finanza pubblica, può anzi tutto rilevarsi come in termini prospettici potrebbe risultare opportuno esplicitare il collegamento tra i saldi inerenti le pubbliche amministrazioni e la gestione del bilancio,

In tal modo, si potrebbe potenziare il rendiconto come strumento complessivo di conoscenza ed analisi della finanza pubblica, facendone un momento di riscontro dell'indirizzo politico-finanziario attraverso la valutazione dei risultati conseguiti. Tale raccordo (con il relativo potenziamento dello strumento del rendiconto) acquisterebbe anche maggiore significatività alla luce della riforma in corso della sessione di bilancio e della riclassificazione del bilancio per programmi e missioni. Infine, una raccomandazione. L'analisi del rendiconto non dà alcuna indicazione sulla qualità della gestione della spesa. Occorrono in futuro indicatori di *performance* sugli obiettivi che diano una valutazione qualitativa della spesa. Occorre dare una dimensione di grande respiro alla stesura del rendiconto, dimensione che l'attuale rendiconto non possiede. Occorre passare da una logica puramente contabilistica ad una sostanzialistica che legga analiticamente flussi di spesa ed obiettivi. Da questo punto di vista, la riclassificazione del bilancio è assolutamente strategica. Vi

l'assestamento di bilancio al nostro esame presenta variazioni di rilevante entità che incidono in misura consistente sui saldi di bilancio, determinando un netto miglioramento dei conti pubblici. Il dato di maggiore rilievo è quello relativo all'aumento delle entrate, stimato in oltre 12 miliardi di euro complessivi, che ha già suscitato un ampio dibattito in Parlamento e nel Paese sia relativamente alle cause che hanno determinato tale importante extragettito che sulla sua destinazione. Anche sul lato della spesa sono state registrate consistenti variazioni che saranno in prosieguo illustrate. L'assestamento, come integrato con l'emendamento approvato in Commissione, contiene quindi l'aggiornamento, ad oltre metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto all'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Come è noto, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto appena illustrato relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene infatti definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto. Più in generale, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate, per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito; per quanto riguarda le spese aventi natura discrezionale, alle esigenze sopravvenute; e per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa) alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Si è rilevata, in passato, ed è stata oggetto di discussione in Commissione e in Aula, l'inadeguatezza dello strumento dell'assestamento quanto meno sotto il profilo della sua collocazione temporale e la sua insufficienza rispetto alle esigenze di controllo degli andamenti della finanza pubblica. Infatti, la non piena disponibilità al 30 giugno, data di presentazione del disegno di legge di assestamento, dei dati relativi all'aggiornamento delle previsioni riguardanti le entrate (ed in particolare l'autoliquidazione delle imposte sui redditi) ha posto il problema relativo all'utilità di mantenere il suddetto termine ultimo del 30 giugno per la presentazione dell'assestamento, considerato anche che l'*iter* viene da tempo concluso in Parlamento durante la sessione di bilancio, come avverrà anche per quest'anno. Si è reso, quindi, necessario aggiornare i dati del disegno di legge originario e ciò è stato effettuato con un emendamento presentato dal Governo in Commissione, che contiene ulteriori rilevanti variazioni sia delle entrate che delle spese ed il cui contenuto richiamerò sinteticamente. I dati contenuti nell'originario disegno di legge di assestamento per il 2007 evidenziano un miglioramento dei saldi di bilancio in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2007. Il saldo netto da finanziare migliora di migliora di 4.165 milioni di euro, pari a circa il 18 per cento rispetto all'entità del medesimo aggregato, indicata dalla legge di bilancio. Il citato emendamento del Governo determina un ulteriore miglioramento del saldo pari ad oltre 7 miliardi di euro rispetto a quello indicato appunto nell'originario disegno di legge di assestamento. Per effetto dei dati contenuti nell'emendamento del Governo, si prevedono infatti maggiori entrate per oltre 12 miliardi di euro, a fronte di minori entrate per circa 7 miliardi di euro, con un saldo attivo quindi di circa 5 miliardi di euro. Per quanto riguarda le spese, viene registrato un aumento di circa 230 milioni, a fronte di una diminuzione pari a circa 2.248 milioni con un saldo positivo quindi pari a circa 2.018 milioni; dato quindi anche questo di grande rilevanza. Tornando al testo iniziale, le maggiori entrate, in linea con il tendenziale a legislazione vigente considerato nel DPEF 2008-2011, sono relative essenzialmente al comparto tributario: si tratta di 7.403 milioni di euro, di euro, 5.038 dei quali relativi alle imposte dirette e 2.365 alle imposte indirette. Le maggiori spese nette derivano principalmente dall'aumento degli oneri di natura corrente al netto degli interessi ma anche, in misura significativa, dalla spesa per interessi (1.365 milioni) e marginalmente dall'aumento degli oneri in conto capitale. Anche in termini di cassa, le previsioni assestate comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA. L'avanzo primario e il risparmio pubblico presentano un netto miglioramento sia in termini di competenza che di cassa. I suindicati dati, quelli cioè recati dall'originario disegno di legge vanno comunque valutati alla luce delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 81 e nella relativa legge di conversione che dispongono la destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2007 alla realizzazione degli obiettivi dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica nonché alla copertura delle rilevanti nuove spese ivi recate. Le risultanze dell'assestamento vanno altresì valutate in rapporto al DPEF 2008-2011 che ha rivisto l'obiettivo di indebitamento netto per il 2007, fissandolo al 2,5 per cento del PIL, che si pone ad un livello inferiore al 2,8 indicato dal DPEF dello scorso anno e confermato dall'aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006), ma superiore dello 0,4 per cento rispetto a quello stimato nell'attuale quadro di finanza pubblica a legislazione vigente, quello cioè stimato al lordo della manovra, di cui al decreto di luglio. Su tali dati si innestano le ulteriori consistenti variazioni, di cui l'emendamento del Governo che determina, come già detto, un *surplus* di risorse per oltre 7 miliardi di euro. L'emendamento è volto, con riferimento alle entrate, ad adeguare le previsioni per il 2007 all'andamento del gettito, anche sulla base dei primi risultati relativi all'autoliquidazione. Nel complesso, si determinano maggiori entrate per 12.122 milioni, a fronte di minori entrate per circa 7.000 milioni, come dicevo, con un saldo netto di circa 5.000 milioni di euro.

riferimento all'IRES, nel dibattito in Commissione, il rappresentante del Governo ha chiarito che l'aumento è riconducibile, per oltre 4.000 milioni, a maggiori versamenti a titolo di acconto che presumibilmente scontano, da parte delle imprese, andamenti ottimistici dell'economia per quanto riguarda i redditi 2007 e un maggiore rigore fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria. Il dato è peraltro destinato a migliorare ulteriormente per effetto dell'aggiornamento delle entrate di settembre, come preannunciato dal Governo in Commissione. Per quanto riguarda invece l'IRE, la forte variazione diminutiva deriva - secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo - da una revisione delle previsioni relative alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, con riferimento in particolare alle pensioni e alle retribuzioni dei dipendenti pubblici, rispetto alle quali la chiusura dei rinnovi contrattuali non si verificherà in tempo utile per generare i riflessi sul gettito fiscale inizialmente stimati. Un altro fattore esplicativo della diminuzione delle previsioni di gettito IRE indicato dal Governo deriva dall'effetto in termini di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi delle spese inerenti agli autoveicoli in relazione alla limitazione della detraibilità delle spese stesse ai fini IVA. Tale spiegazione, in verità, non è risultata del tutto convincente (ne abbiamo discusso in Commissione), stante la rilevante entità (oltre 4.000 milioni di euro) del minor gettito IRE rispetto all'aumento previsto nel disegno di legge originario (di oltre 3.000 milioni di euro), che riflette evidentemente un fenomeno di più estesa consistenza. Altre variazioni significative riguardano le imposte sostitutive, in un aumento per oltre 2.000 milioni di euro: l'IVA, con un incremento di oltre 2.700 milioni di euro;

in diminuzione di circa 2.000 milioni di euro. In particolare, vi è una flessione per 1.300 milioni di euro dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativa alle risorse proprie dell'Unione Europea, conseguente alla rideterminazione delle quote richieste dalla Commissione quale contributo al bilancio comunitario per il corrente anno. Anche su tale variazione occorrerebbe un supplemento di valutazione poiché, ove essa fosse di carattere permanente, legata cioè alla riduzione della contribuzioni al bilancio UE conseguente alla ridefinizione delle prospettive finanziarie 2007-2013, si determinerebbe un ulteriore rilevante miglioramento dei nostri conti pubblici. Nel medesimo stato di previsione un'altra variazione importante riguarda la riduzione di 750 milioni del servizio del gioco del lotto, per adeguare lo stanziamento al prevedibile andamento del gioco stesso. Nel rinviare, per il resto, al testo del disegno di legge e degli emendamenti, in particolare a quello del Governo, provo a trarre qualche conclusione e valutazione politica. va evidenziato che il cospicuo extragettito rilevato, oltre ad incidere positivamente sui conti pubblici, determina le condizioni per un'attenuazione della pressione fiscale senza mettere in discussione gli obiettivi di finanza pubblica fissati nel DPEF. Vanno certamente approfondite le ragioni che hanno determinato le maggiori entrate rilevate, anche per misurarne la parte strutturale, ma è già possibile affermare ragionevolmente che probabilmente esse scaturiscono da concause riconducibili ad un più virtuoso comportamento dei contribuenti, ai primi risultati delle misure di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, al favorevole andamento del ciclo economico e ad altre cause più specifiche, come ad esempio gli effetti delle misure conseguenti alla sentenza IVA sulle automobili. Su tali elementi si chiede al Governo di fornire maggiori informazioni in futuro anche per meglio valutare l'impatto dell'andamento del gettito sulle previsioni che saranno fissate nella prossima legge finanziaria. è opportuno rilevare che l'andamento positivo della finanza pubblica, registrato con l'assestamento, si pone in evidente controtendenza con i risultati in corso d'esercizio rilevati in quasi tutti gli anni passati, allorquando si è dovuto spesso fare ricorso a manovre correttive per far fronte al peggiore andamento dei conti pubblici che veniva riscontrato. Si tratta, quindi, di un netto miglioramento nella gestione della finanza pubblica destinato a produrre effetti importanti, oltre che sui conti pubblici, anche sulle famiglie e sull'economia che, mi auguro, si produrranno, con le misure delineate nella risoluzione parlamentare relativa al DPEF, già con la prossima manovra finanziaria.

del suddetto decreto-legge n. 81 dello scorso luglio. Tale invarianza dei dati fondamentali di finanza pubblica fa presupporre che l'ulteriore extragettito rilevato con l'emendamento del Governo sarà, in tutto o in parte, probabilmente utilizzato nel contesto degli strumenti per la manovra di bilancio preannunciati dal Governo, tra i quali è previsto un decreto-legge coevo al varo della legge finanziaria destinato ad anticipare alcuni degli impegni sottoscritti dal Governo. L'auspicio è che tale decreto, ove dovesse essere coperto con le risorse che oggi registriamo in aumento, si indirizzi verso l'inizio della restituzione delle imposte ai contribuenti ed eventualmente alla realizzazione di infrastrutture. Il contenuto complessivo dell'assestamento costituisce, quindi, un tassello importante della manovra che sarà varata dal Governo nei prossimi giorni e i cui obiettivi fondamentali sono già stati indicati dal Ministro dell'economia nell'audizione di ieri conformemente al DPEF e alla relativa risoluzione parlamentare. Per le ragioni che ho illustrato e per quelle contenute nella relazione scritta depositata, invito l'Aula del Senato ad approvare il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e gli emendamenti già approvati in Commissione.

nella relazione del senatore Legnini. È la seconda volta nel corso del 2007 che registriamo un extragettito: il primo era pari a 7,4 miliardi,

di marzo e certamente inferiore al 3 per cento che è il livello previsto dal Patto di stabilità. Quindi, il nostro Paese è assolutamente in regola. I conti cominciano ad essere in ordine. Ci sono circa cinque miliardi in più che devono essere registrati e che sono il risultato della somma algebrica tra la riduzione di 4,2 miliardi dell'IRE

alto rispetto alle previsioni di spesa e di entrata. Credo che la risposta che il Governo ha fornito in Commissione sia soddisfacente: le previsioni solitamente non possono valutare correttamente e fino in fondo i flussi dei dati dell'autoliquidazione e, inoltre, le entrate del primo mese preso in considerazione, cioè del mese di gennaio, sono generalmente poco riproducibili sul piano statistico, perché dipendono ovviamente da come si chiude il mese di dicembre, cioè l'anno precedente. Allora, è proprio l'assestamento e, in questo caso, l'emendamento del Governo che accerta e adegua le previsioni di entrata e di spesa. Per quanto riguarda lo scostamento relativo all'IVA, il Governo ha affermato che nei primi otto mesi non c'è stato un ricorso generalizzato alla deducibilità dell'IVA sulle auto aziendali.

diminuita rispetto a quanto si è accertato con l'assestamento. Più nel dettaglio, è interessante notare che flette l'IVA

Le origini dell'extragettito, come sappiamo, sono dovute all'andamento del ciclo e una buona parte di esso è dovuto anche al contrasto all'evasione fiscale che sta modificando il rapporto tra i contribuenti e l'amministrazione fiscale. Questa parte strutturale può essere certamente utilizzata per una riduzione del carico fiscale in generale; decideremo nei decideremo nei prossimi giorni se nei confronti del sistema delle imprese, dei redditi più bassi o dei lavoratori. Credo che comunque la questione di fondo sia questa: la parte strutturale può essere utilizzata per ridurre la pressione fiscale. In particolare, ritengo che l'incremento dell'IRES, che si è verificato in misura importante,

emerge base imponibile, in particolare, relativa a tasse e contributi inizialmente evasi. L'assestamento, tra l'altro, deve aggiornare le previsioni e probabilmente la riduzione che si è verificata dell'IRE dovrebbe essere correlata, a mio avviso, alle restituzioni intervenute nel 2007, cioè agli effetti della finanziaria del 2007, in particolare, alla restituzione del cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti. In altre parole, la politica fiscale avviata lo scorso anno sembra esplicare gli effetti redistributivi in misura maggiore rispetto a quanto era stato previsto. E, se c'è da fare una critica al Governo e, diciamo, a tutta la maggioranza, è che forse dovevamo spiegare meglio il tipo di processo redistributivo che abbiamo iniziato con la scorsa finanziaria. Infine,

Anche su questo aspetto sarebbe interessante conoscere quanta è la parte strutturale di queste minori spese: infatti, se ci fosse una parte strutturale significativa, certamente anch'essa potrebbe essere utilizzata

obiettivamente, l'extragettito produce un aumento del carico fiscale - questo è ovvio - e io credo che sia necessario intervenire, attraverso l'utilizzo dell'extragettito, per ridurre le tasse e portare almeno

necessità o meno di ridurla: credo che dobbiamo solo applicare la legge, la quale già prevede che le maggiori entrate, eccedenti rispetto alle previsioni e di carattere strutturale, debbano essere indirizzate a ridurre la pressione fiscale. Credo, mi auguro e chiedo al Governo che quest'operazione venga compiuta con la prossima finanziaria. *(Applausi

rilevato dall'ECOFIN, quindi, le entrate sono aumentate di 4.165 milioni, al netto delle maggiori spese, quindi, un saldo da finanziare nella misura del 18 E, anche qui, il gioco delle tre carte ha funzionato bene: "il tesoretto" non c'era, il saldo non c'era (per cui il collega Baldassarri, che ha sempre parlato di falso in bilancio, è stato sbeffeggiato più volte), arrivava il vice ministro Visco a dire che non lo sapeva, ma in realtà sappiamo tutti com'è andata.

È una contabilità creativa che fa impallidire quello che pensate di Tremonti: qui siamo al gioco delle tre carte dei tre bari di Napoli (e non solo di Napoli, ovviamente), che le mescolano per motivi politici.

di questi 29 miliardi. Il resto dov'è andato? È andato da altre parti, con un aumento della pubblica amministrazione, in qualche rinnovo contrattuale sicuramente al di sopra del tasso di inflazione, ma soprattutto

l'aumento delle tasse, di cui gli italiani si sono ben accorti, questo è evidente. Non solo, ma ad aggravare la situazione, ci sono gli aumenti delle spese della pubblica amministrazione. Avete dovuto correggere i risparmi dei Ministeri prevedendo una deroga prevedendo una deroga per l'anno 2007, introdotta con l'articolo 7, sulla contrazione della spesa corrente dei Ministeri mediante accantonamenti. Anche per questo avremo maggiori spese. Avete detto che l'Italia era ripartita, che c'erano questi grandi successi. Appena vi hanno visto, sono aumentate le tasse. Beh, certo, quando uno incontra i briganti, la prima cosa che sente

magra, forse di soli 10 miliardi. Ebbene, intanto iniziamo a dire che i costi della pubblica amministrazione - l'avete già detto, l'ha detto il Ministro - si assestano sui 25 miliardi,

incattiviti per scelta ideologica. Signor Presidente, sottolineo che era difficile raggiungere tre obiettivi contemporaneamente. l'aumento delle tasse, che avete fatto tranquillamente, pur avendo il "tesoretto". In periodi difficili, la Casa delle Libertà è riuscita a ridurre

avevate i sindacati pronti al tavolo, disarmati, in pace: erano lì con le colombe, con fiaschi di vino e quant'altro. Li avevate tutti.

i funzionari li avevate: nei nodi importanti del Paese siedono persone vicine a voi. Avete mandato via mezza classe dirigente a spese di Pantalone, con cifre di 30 milioni di euro, per poter avere persone fidate. Avete aumentato la spesa pubblica. Ma

Partiamo da un single, che ha un reddito di 20.000 euro: un buon operaio con straordinari. Bene, già non ci arrivava prima: spese essenziali 16.000 euro, necessarie 6.414, lasciamo perdere le voluttuarie, arriviamo a circa

ammontano a 870 euro; ha avuto un aumento dell'incidenza del costo della vita, nel giro di un anno del vostro Governo - certo, vostro Governo: se vi prendete tutti i meriti, prendetevi anche questa situazione del Paese - del 5,56

29.000 euro. Vi ricordo che il presidente del Consiglio, Romano Prodi, aveva promesso, prima del *Family Day*, di destinare tutto il "tesoretto" alle famiglie.

al diciassettesimo giorno; prima arrivava al diciottesimo. Con il terribile Governo Berlusconi arrivava a due giorni in più, ora campa due giorni in meno. Forse, per i ricchi qualcosa di meglio c'è stato,

ci meravigliamo perché c'è un comico che vuol fare politica, ma abbiamo un politico che è un ottimo comico e si chiama Romano Prodi. *(Applausi

che assumono un ruolo rilevante in un corretto funzionamento della democrazia parlamentare per verificare lo schema di previsione di entrata e di autorizzazione di spesa. I relatori hanno edulcorato però il loro giudizio, non hanno recepito quello che invece c'era di più profondo in alcune critiche da parte della Corte dei conti. Siamo lontani da una riforma del bilancio come momento non di riclassificazione contabile ma di una strategia di razionalizzazione finanziaria amministrativa. Vogliamo, onorevole Sottosegretario, la realizzazione compiuta del Sistema lei non ci ha dato nessuna risposta in Commissione, lei dovrebbe dirci chi rema contro il completamento di un progetto che dà immediatamente al centro, all'organo di governo, la possibilità di verificare l'andamento dei flussi di finanza pubblica. L'articolazione delle funzioni obiettivo necessiterebbe dell'introduzione di indicatori di prodotto e di impatto all'interno delle note preliminari di bilancio coerenti con le direttive generali. Quello che manca è la possibilità di una valutazione economico-finanziaria delle risultanti di entrata e di spesa in relazione ad obiettivi stabiliti dagli indicatori di efficacia e di efficienza e il raccordo tra i dati di bilancio e i dati dei conti delle pubbliche amministrazioni. Sul piano dei saldi differenziali, l'indebitamento certificato al 2,4 per cento al netto della sentenza UE sulla indetraibilità dell'IVA e per l'accollo dei debiti connessi alla TAV è un dato inoppugnabile rispetto alla tanta demagogia: altro che *due diligence* di *deficit* al 5 Altro dato positivo è quello relativo al ricorso al mercato, che si cifra a 150.671 milioni di euro, che non è stato influenzato dalle vostre scelte, perché è stato abbattuto da scelte precedenti. Va sottolineato il dato evolutivo negativo del debito degli enti locali, cresciuto del 20 per cento, corrispondente ad 1,3 punti del PIL. Volete acquisire anche questo dato, per cortesia? Sul piano dei risultati di gestione, emerge la crescita rilevante delle entrate tributarie ed extratributarie. Ma il dato più rilevante Ma il dato più rilevante del conto di bilancio è rappresentato dal sensibile incremento delle eccedenze di spesa registrate nei vari stati di previsione invertendo il *trend* di diminuzione del periodo 2002-2005. Si tratta di una vera e propria patologia, sia programmatica che gestionale del sistema, in quanto tali eccedenze costituiscono un insieme di atti di impegno e di pagamento superiori alle cifre stanziate nel bilancio di previsione determinate una sanatoria *ex post* con l'articolo 7 del disegno di legge. È una vera e propria violazione di legge, su cui l'organo di controllo non esprime un giudizio di correttezza. rappresentano una grave anomalia rispetto all'esercizio concluso: stiamo parlando di 4 miliardi in termini di competenza e in tale azione si sono distinti il Ministero dell'istruzione e quello delle infrastrutture. Per quanto riguarda poi il rendiconto dell'entrata, la Corte dei conti ha segnalato molte incongruenze contabili e anomalie interne al rendiconto, come l'emergere di una serie di voci di bilancio classificabili come insussistenze attive e passive, vere e proprie discordanze tra i relativi importi con quelli risultati dalla contabilità delle amministrazioni. La Corte dei conti ha mancato la certificazione di regolarità al capitolo 7060, relativo al Ministero delle infrastrutture, a fronte delle discrasie emerse tra i pagamenti disposti a valere delle disponibilità del Fondo opere strategiche per cui non vi sarebbe stata la dovuta scritturazione in contabilità finanziaria. Vi sarebbero state anticipazioni che non hanno trovato sistemazione dentro la chiusura dell'esercizio. discordanze tra gestione del bilancio e quella di tesoreria comprese nel conto del patrimonio in relazione ai conti correnti, agli incassi da regolare e alle altre gestioni per la passività finanziaria, incongruenze sulla disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria sui pagamenti da regolare sul conto dare e avere nell'ambito del servizio di tesoreria centrale e provinciale. Si registrano mancanza e incompletezza della documentazione giustificativa sulle variazioni intervenute sulle attività finanziaria e non finanziaria. Emerge dunque un quadro allarmante per quanto attiene i documenti contabili. Il relatore Battaglia ha edulcorato il giudizio della Corte dei conti. Per quanto riguarda l'assestamento siamo in presenza solo di un rispetto formale del documento contabile e non sostanziale con evidenti valutazioni sulla tempistica del provvedimento. di legge *ab origine* presentava previsioni di entrata che non tengono conto degli effetti dell'autoliquidazione delle imposte sui redditi, il che da luogo alla presentazione di emendamenti che tengono conto, da parte del Governo, delle più aggiornate previsioni di gettito. Ogni giorno spuntano nuovi tesoretti: è stato presentato un emendamento in Commissione bilancio per 7 miliardi di euro, mi auguro che gli emendamenti non siano terminati e che non ne venga presentato uno ulteriore, magari con Ma qual è la per cifra vera da mettere nel bilancio di assestamento? Perché procedete in modo così distorto? Perché volete spendere questo tesoretto con nuova spesa che accontenti i componenti della vostra vostra coalizione, così eterogenea, e che va aumentando giorno dopo giorno? Abbiamo espresso molti interrogativi in Commissione. Non abbiamo trovato risposta. Un primo problema emerge, per esempio, dalla maggiore spesa per interessi, gran parte ricondotta ai maggiori interessi da corrispondere sui conti correnti di tesoreria intestati a soggetti pubblici e privati. Fa presumere un aumento delle disponibilità medie detenute dai soggetti pubblici e privati. È forse inopportuno, onorevole sottosegretario, che il Parlamento conosca le cause di variazione delle giacenze e l'indicazione degli enti intestatari dei conti variati? (*Segue* EUFEMI). Mi auguro che nella sua replica ci sia una risposta. Si registra l'assenza di effetti in termini di competenza economica. Sono necessarie integrazioni sulla dinamica di spesa non in linea con l'andamento incrementale dei tassi di interesse di mercato. Si registrano operazioni di pronti contro termine senza alcuna variazione compensativa. E veniamo alle variazioni di entrata. L'IVA non sconta l'autorizzazione UE a limitare al 40 per cento il diritto all'esenzione IVA detraibile, su questo si è soffermato anche il relatore, mi auguro che lui abbia più fortuna. Nell'atto 1485 prevedevate 4.600 milioni di euro in termini di competenza e 2.300 per cassa: richiederebbe un assestamento del maggior gettito. chiarimenti in ordine ai Tabacchi, al Lotto e ad altre attività e un chiarimento rispetto alle regolazioni debitorie ASL, indicate, solo per cassa, in 3.186 milioni. Come mai non si riflette anche sulla competenza, invece, l'importo autorizzato di 3.000? Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con la manovra emendativa voi non fate un'operazione di trasparenza dei conti pubblici ma utilizzate le maggiori entrate per anticipare la finanziaria nascondendo il quadro di finanza pubblica e questo non è consentito dalle norme sulla contabilità di Stato. Voi state nascondendo i conti pubblici perché fate una manovra con l'assestamento, poi ne fate un'altra con il decreto, poi ne fate un'altra ancora con la finanziaria che poi la chiamerete snella perché non volete spaventare gli italiani. Ma gli italiani non sono così stupidi, onorevole rappresentante del Governo. Voi state alimentando il fenomeno delle «variazioni postume». Volete fare una finanziaria *bis* utilizzando lo strumento dell'assestamento, e i tanti rigoristi che cosa dicono rispetto a queste anomalie? La sottostima delle entrate 2007 ha già inficiato la veridicità della decisione di bilancio, vanificando il potere parlamentare di assumere decisioni in ordine alla destinazione delle risorse disponibili in un quadro chiaro, coerente e non alterato, confuso, incoerente e contraddittorio come voi state facendo. Voi state agendo nel senso di non rendere conoscibili e governabili gli andamenti dei grandi aggregati di bilancio, non esiste al mondo che si possa controllare la spesa senza *budget*. La funzione dell'assestamento è quella di correggere gli andamenti divergenti e la base informativa della Corte dei conti è stata in grado di orientare le nostre scelte ed i nostri giudizi. Non viene evitato l'aggiustamento delle autorizzazioni. Vi è un'evidente forzatura in questo senso e il senatore Calderoli ha presentato un ordine del giorno che io condivido pienamente perché quelli che state operando non sono interventi marginali. Diventa una finanziaria infrannuale per svuotare quella vera. Dovremmo invece guardare al consolidamento della cornice finanziaria, perciò non dovrebbero subire peggioramenti il livello del ricorso al mercato (come invece avviene per l'1,1 per cento, e risulta incrementato di 2 miliardi di euro) e i primi due titoli della spesa; il che significa più debito e più costo per il servizio dello stesso. Tale debito è cresciuto sotto la vostra gestione di 42 miliardi di euro in valore assoluto (mese su mese, da maggio a maggio). Questa è la vostra *mala gestio*: aumentano le autorizzazioni finali per 1,5 miliardi, crescono le spese correnti nei trasferimenti agli enti locali per 2,2 miliardi, interessi per 1,5 miliardi e un fondo autorizzazione di cassa per 1,5 miliardi. Evitate allora di fare ulteriori danni! Vi abbiamo dimostrato che con la vostra finanziaria la linea della povertà; non possiamo allora esprimere un giudizio che non sia allarmato sul *trend* delle vostre scelte, in particolare

pertanto, avete bisogno di colpire l'immaginario collettivo con i Valentino Rossi, come avevate fatto 10 anni fa con il povero Pavarotti, costretto a recarsi nello studio del ministro Turco a mendicare una sanatoria. Questo avete voluto e questo vorreste che facesse anche Valentino Rossi. Come dicevo, colpite l'immaginario collettivo con il grande evasore

introducendo il conflitto d'interessi, pertanto esprimiamo un giudizio preoccupato, perché con queste scelte non si opera il consolidamento dei conti pubblici, non si va verso l'abbattimento del debito pubblico - la vera palla al piede dell'economia - né verso un contenimento della spesa pubblica, ma in tutt'altra direzione. Onorevole Sottosegretario, ho avuto la determinazione e la costanza di chiedere in questi giorni il bollettino mensile delle entrate fiscali che abbiamo avuto soltanto questa mattina. Tale bollettino dovrebbe essere a disposizione del Parlamento e il vice ministro Visco aveva assicurato che sarebbe stato disponibile il dieci di ogni mese

erano già state operate con la precedente decisione di bilancio. Proprio quel *trend* di crescita delle entrate sta a dimostrare che avete colpito con le addizionali cresciute del 10 per cento, quelle comunali del 30 per cento). Quella è la dimostrazione che avete torchiato gli italiani! Per queste ragioni, signor Presidente, credo che da parte mia non ci possa essere consenso

*(AN)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ricordo che nel dicembre del 2006, al momento di discutere la finanziaria per il 2007, denunciai in quest'Aula il falso in bilancio che il Governo stava commettendo e la sua maggioranza parlamentare stava approvando.

una soddisfazione, perché anche per questo Governo due più due deve fare quattro; amara, perché si conferma che da dieci mesi la Repubblica italiana opera con un bilancio falso, che neanche questo assestamento di bilancio correggerà. Signor Presidente, i numeri sono i seguenti: a dicembre potete ricorrere ai resoconti parlamentari, cari colleghi - il Governo e voi della maggioranza avete approvato un numero: 703 miliardi di euro di gettito previsto per il 2007. Questo numero era falso e sottostimato per ben 23 miliardi di euro: si sarebbe dovuto scrivere 726 miliardi di euro marzo 2007, il Governo, nella Relazione unificata, porta i 703 miliardi di dicembre a 713 miliardi e inventa il tesoretto n. 1. Nel giugno 2007, nel DPEF il Governo porta quel numero a 715,4 e inventa il tesoretto n. 2. Il 5 luglio 2007, il Vice ministro dell'economia dichiara che quel numero è diventato 717 miliardi e si inventa il tesoretto n. 3. A fine agosto 2007, il Governo comunica ufficialmente al Paese che l'andamento del gettito 2007 si rapporta a 720 miliardi di euro:

che quell'importo si rapporta ad altri 7od 8 miliardi in più: 728 miliardi di euro. Bene, lanciai una scommessa in quest'Aula: ho vinto la scommessa. Cari colleghi della maggioranza, se aveste accettato quella scommessa, oggi dovreste pagare una cena a tutti i colleghi del Senato, ovviamente non a carico del bilancio pubblico. Signor Presidente, è una constatazione molto amara, perché bastava fare due moltiplicazioni e un'addizione per avere a dicembre la verità. Molto amara per voi della maggioranza perché, se aveste costretto il vostro Governo a dire la verità con 23 o 24 miliardi di euro in più di gettito disponibile a dicembre, avreste potuto rapportare a meno dell'1 per cento il *deficit* pubblico oppure realizzare provvedimenti utili per la collettività. Entro quell'importo di falso in bilancio poteva rientrare un forte sgravio fiscale alle famiglie e non - come i dati pubblicati oggi dal quotidiano «il Giornale» dimostrano - un appesantimento, una forte riduzione del potere di acquisto proprio per le famiglie a reddito medio e medio basso. Poteva rientrarci l'azzeramento dell'ICI sulla prima casa; poteva rientrarci il dimezzamento dell'IRAP per le piccole e medie imprese. voi della maggioranza - avete rinunciato a provvedimenti di questa portata per seguire pedissequamente un falso in bilancio prodotto dal vostro Governo.

Ma veniamo al provvedimento di oggi, signor Presidente. Qui nascono, da ieri sera, in sede di audizione del Ministro dell'economia, a questa mattina in Aula, alcuni enormi misteri

come mai, avendo il Governo dichiarato che c'è un extragettito, che vi

che quest'Aula è chiamata ad approvare, il Governo ne ha indicati solo 12? Dove sono gli altri 13 miliardi dichiarati dal Governo non dal senatore Baldassarri, perché il senatore Baldassarri la dichiarazione l'aveva fatta a dicembre, il Governo l'ha fatta a settembre 2007)? Perché nell'assestamento si occultano ancora oggi 13 miliardi? E non mi si venga a rispondere che stiamo parlando del bilancio dello Stato, mentre i numeri che ho citato fanno riferimento al bilancio consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni. Qui parliamo di gettito erariale, il gettito erariale è scritto con lo stesso importo sia nel bilancio dello Stato, sia nel bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni. Vorrei davvero che l'Aula avesse la possibilità - lo dico anche per i colleghi della maggioranza - di avere una risposta su questo mistero. Il secondo mistero è quello che emerge anche dall'intervento del collega Legnini. Se con questo assestamento il Governo porta a gettito 12 miliardi di euro in più, delle due l'una: o parallelamente si riduce l'obiettivo di *deficit* pubblico, oppure vuol dire che si stanno nascondendo pari importi di spesa. Il mistero, cari colleghi, è che il Governo viene qui a nascondere il totale del gettito, lo mette parzialmente nell'assestamento per 12 miliardi, e i saldi finanziari non cambiano di mezzo euro. Anzi, nel DPEF, con questo enorme extragettito, il Governo ha detto e scritto che quest'anno avremmo avuto un *deficit* del 2,1 per cento: ora però ha deciso di aumentarlo al 2,5 Questo è il mistero. C'è una valanga di entrate in più, però il *deficit* non solo non diminuisce aritmeticamente, ma aumenta: perché? Perché si sta nascondendo, oltre al gettito, anche l'imponente aumento di spesa corrente che emergerà solo a consuntivo nel 2007, forse quando avremo i consuntivi, nella primavera del 2008. terza riflessione, signor Presidente: questo assestamento rappresenta un forte indizio che il Governo intende reiterare il reato di falso in bilancio sul 2008 perché, mettendo solo parzialmente il gettito nel bilancio 2007, consentirà tra qualche giorno - e lo verificheremo - una stima di gettito preventivo per il 2008 anch'essa largamente sottostimata.

falsificando il dato tendenziale e dicendo poi che il gettito effettivo è più alto; ecco quindi un extragettito. Aspettiamoci una serie di tesoretti anche per l'anno 2008.

Colleghi della maggioranza, che vi vedo leggendo i giornali, litigare l'un l'altro discutendo se aumentare di 82 centesimi al giorno le pensioni minime della gente che veramente non arriva neanche alla terza settimana, guardate i dati che pubblica oggi "il Giornale", fate le vostre valutazioni indipendenti. Ma se è vero che ci avete accusato, durante i cinque anni del Governo Berlusconi, di aver affamato gli italiani, che non arrivavano alla quarta settimana, ebbene, se ciò è vero, è altrettanto vero, sulla base dei dati 2007, gli italiani non arrivano alla terza settimana. Signor Presidente, ho presentato un emendamento che in Commissione è stato giudicato inammissibile perché si dice, con il solito sofisma giuridico, che l'assestamento di bilancio è una norma di forma non può incorporare provvedimenti di sostanza. Siamo al paradosso, ad una situazione kafkiana! Ha ragione il collega Legnini a dire che siamo di fronte ad un assestamento di bilancio gigantesco,

Qui i numeri del Governo avrebbero richiesto un assestamento di 24-25 miliardi che il Governo limita, nascondendo una parte, a 12 miliardi. Ma è pur sempre un assestamento di 12 miliardi di euro, 24.000 miliardi di vecchie lire. E questo lo chiamiamo aggiustamento di forma. Allora, insisto in Aula su un emendamento molto semplice. Vorrei che vi riflettessero i colleghi della maggioranza, soprattutto quelli che, almeno a parole, si dicono più vicini alle esigenze della parte più bisognosa della nostra popolazione. L'emendamento avanza le seguenti semplici proposte: voi avete disperso, a fine luglio, con il decreto chiamato da voi tesoretto, 7 miliardi di spesa pubblica, dei quali 900 milioni sono stati dedicati all'aumento delle pensioni minime, cioè 82 centesimi al giorno.

utilizziamo quei 7 miliardi che avete sperperato nei bilanci dei vari Ministri, sotto voci pseudosociali,

Sarebbero 4,3 miliardi dei 7 che voi avete già speso e che sarebbero recuperabili, abrogando quel decreto che avete trasformato in legge. per la differenza, fino alla concorrenza dei 7 miliardi di euro, l'azzeramento dell'ICI sulla prima casa per tutti, che costa 2,3 miliardi Se fate la somma sono 6,8 miliardi, esattamente l'importo che avete sperperato senza copertura a luglio-agosto, perché non c'era ancora l'assestamento di bilancio e avete detto che la copertura era a futura memoria, cioè con l'assestamento che stiamo discutendo adesso. Quindi, avete fatto passare un decreto-legge privo di copertura finanziaria, dicendo che sarebbe stato coperto con l'assestamento. Allora, l'emendamento che ho presentato a mia firma contiene una semplice usiamo una parte di quello che voi chiamate extragettito, senza toccare gli equilibri di finanza pubblica (operazione che io chiamo falso in bilancio, superiamo anche questa diatriba, adesso i soldi ci sono,

gioco delle tre carte e spesa messa nelle mani e nei portafogli, a discrezione dei Ministri e dispersa automaticamente come dimostra, signor Presidente, questo assestamento: un aumento di entrate di 12 miliardi, che non fa ridurre di un euro il*deficit,* perché evidentemente il Governo sa che quelle maggiori entrate se le è già spese se le è già spese e continuerà a spenderle con i prossimi provvedimenti. Non credo però sia tollerabile, e concludo, signor Presidente, che si reiteri il reato. Voglio avvertire l'Aula sin da questo momento che se il Governo,

aggiornato alla crescita del prodotto interno lordo, che purtroppo sarà molto minore di quanto il Governo ha previsto come obiettivo, moltiplicato il rapporto entrate-PIL (l'elasticità 1,1 dichiarata nei documenti ufficiali del Governo), se il numero che apparirà per il 2008 corrisponderà a questi criteri, ebbene, signor Presidente, cari colleghi, saremo al secondo reato consecutivo di falso in bilancio. Lo chiamerete poi recupero con la lotta all'evasione; potrete chiamarlo Pippo, Pluto o Paperino

Francamente continuo a non capire perché la Corte dei conti, alta magistratura contabile, e la Presidenza della Repubblica, più alta magistratura dello Stato, di fronte a tali valutazioni, rispondano con un silenzio che è incomprensibile. Delle due l'una: o sto dicendo cose folli, oppure ho ragione. La stessa cosa è avvenuta a dicembre

*(FI)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi,

attenta agli effetti della finanza pubblica e al contenimento soprattutto della spesa, siano proprio null'altro che favole belle. Infatti, se consideriamo, ad esempio, l'incremento delle spese notiamo che la spesa corrente nel suo complesso è aumentata del 2,9 per cento, ben al di sopra

A fronte di tali crescite si registrano trasferimenti complessivi all'amministrazione pubblica, quindi spese di funzionamento soprattutto di Province, Comuni e Regioni, nell'ordine del 5-6

in evidenza l'aumento sostanziale della spesa e avete in qualche modo quadrato il bilancio, grazie anche all'andamento positivo delle entrate. Questo è il tema che riguarda principalmente l'assestamento

non era mai capitato di assistere ad un Governo così schizofrenico che durante l'estate 2006 afferma che la situazione economica è peggiore di quella del 1992,

tesoretto e far crescere gli appetiti della multiforme compagine che lo compone affinché ciascuno potesse reclamarne una spoglia, un brandello.

spesso improduttiva e dannosa. Basta leggere l'editoriale di oggi del «Corriere della sera» per rendersi conto di come la vostra spesa va a favore non della parte debole della popolazione, ma di quella sindacalizzata. il recente accordo sul *welfare* vede un miglioramento delle condizioni pensionistiche dei lavoratori sindacalizzati a buon livello di reddito, aumentando i contributi per i non sindacalizzati, per quelli che stanno fuori del mercato del lavoro; il che, ovviamente,

Il tutto senza risolvere un piccolo problema: la crisi economica che deriva dalla crisi del *subprime*, che è iniziata negli Stati Uniti e poi si è diffusa in tutta Europa. Bene, tutti gli organismi di ricerca, ma anche lo stesso Governo, ammettono che già nel 2007 ci sarà una diminuzione della crescita del prodotto interno lordo in conseguenza di quell'evento la diminuzione della crescita del prodotto interno lordo non potrà non riflettersi anche nel rapporto *deficit*-PIL; obiettivo del rapporto *deficit*-PIL, tuttavia, come ha chiarito ieri il Ministro dell'economia e delle presso le Camere, resta il 2,5 per cento. Tuttavia, questo 2,5 per cento non può essere più mantenuto dopo che sono cambiati i fondamentali dell'economia. Quindi, qualcosa andrebbe fatto per migliorare già i saldi del 2007; nulla si fa, anzi, emerge un ulteriore tesoretto che non vorrei, signor Presidente, il Governo avesse intenzione di spendere già nel corso dell'anno per soddisfare qualche appetito che, a questo punto, non si può definire altro che pre-elettorale da parte della maggioranza di Governo. Non dimentichiamo che ai sensi, non solo della legge di contabilità, ma soprattutto del buon senso, non è pensabile spendere le maggiori entrate che non derivano da variazioni normative, ma dall'andamento spontaneo delle entrate, per finanziare nuove spese. Quindi, se ci sono maggiori entrate, queste vanno conservate

non è più quello originario prefissato nel DPEF, anzi, c'è chi inizia a temere che vada pericolosamente vicino al 3 per cento. Quindi, vedremo poi, in costanza di un'ulteriore diminuzione del prodotto interno lordo

Certo, qualche preoccupazione ci resta se la manovra con la finanziaria ha l'entità che è stata preannunciata dal Ministro dell'economia e delle finanze, cioè circa dieci miliardi al netto - perché al netto sembra essere - dell'eventuale manovra che si farà in materia di *welfare*; se anche quella, che dovrebbe finire in un collegato e non direttamente nella finanziaria, si sommerà alla manovra con la finanziaria, restano da capire gli effetti economici di carattere depressivo che questa manovra avrà e, secondariamente - cosa assolutamente non banale - come si coprirà. Credo, infatti, che sia molto difficile che si possa coprire una manovra dell'ordine di almeno 15 miliardi di euro, 30.000 miliardi delle vecchie lire, semplicemente facendo ricorso a immaginifici contenimenti della spesa. Se dobbiamo, anche in questo caso, trarre insegnamento da quello che ci ha detto ieri il Ministro dell'economia davanti alla richiesta di tagliare la spesa a tutti i Ministeri sono arrivate offerte di tagli reali nell'ordine di un miliardo di euro, a fronte di richieste di incremento della spesa dell'ordine di 20-30 miliardi. *(Applausi dal Gruppo* *FI).* Probabilmente, andrà a finire che o non si farà assolutamente niente o si aumenteranno le tasse, cosa che temo perché probabilmente 6 miliardi di rettifica alle entrate, che non sono altro che un aumento delle tasse nominali, si farà in finanziaria, o, se in qualche modo taroccheranno i dati per far finta che non succeda niente, sperando che in questo modo, con l'avvelenamento dei pozzi, la maggioranza che subentrerà l'anno prossimo a questo Governo fallimentare, si assuma la responsabilità di risolvere il problema.

negli anni scorsi, è aumentata la base contributiva in costanza di diminuzione di aliquote nominali. Si è fatto in Italia con il precedente Governo quello che è stato fatto in molti Paesi europei: abbassando le aliquote nominali, si è allargata la base e aumentato il gettito, e questo è un risultato tangibile. L'altro risultato deriva dal fatto che nel 2006, con il decreto estivo, furono introdotte misure, benevoli, potremmo definire alquanto forti, sulla tassazione del reddito dell'impresa, trasformando, per esempio, molti costi in reddito, e quindi tassandoli, in qualche modo spremendo le imprese, tanto che molte di esse probabilmente non saranno in grado di mantenere la propria attività a lungo in modo fruttuoso. Si è però fatto però fatto rinvio, da parte del Governo o, più precisamente, dal Vice Ministro che si dedica ai problemi fiscali, ad una figura retorica, la cosiddetta *fiscal compliance*. Ovviamente, quando si deve dire una cosa banale, non si parla mai in italiano ma si suole far riferimento ad una lingua straniera; la potremmo tradurre in qualche modo con l'espressione - se mi è consentita - di "strizza fiscale". Entrato, cioè, in funzione il nuovo Governo, i contribuenti si sarebbero impauriti, decidendo spontaneamente di andare a portare i loro soldi alla sede del Tesoro. È ovvio che si tratta di un comportamento poco credibile, ma finché restiamo nell'impostazione dei presupposti intellettuali, ci si potrebbe anche stare; l'emendamento, presentato dal Governo e approvato ieri dalla Commissione bilancio, dimostra espressamente che la questione della *fiscal compliance* è una vera e propria bufala. se consideriamo - e basta guardare le carte - la tabella delle entrate, com'è stata riscritta dal Ministero dell'economia, vediamo che a titolo di IRE (e cioè la vecchia IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche) abbiamo una riduzione di oltre 4 miliardi. riduzione di oltre 4 miliardi. Questa, sommata algebricamente all'aumento di 3 miliardi presente nel testo dell'assestamento, fa sì che, rispetto alla legge di bilancio, vi sia una diminuzione netta di oltre un miliardo di euro. Tra l'altro tra parentesi, questa diminuzione viene riferita alle ritenute dei lavoratori dipendenti. Ciò vuol dire che a livello di IRPEF - e il Governo non ne ha assolutamente spiegato bene i motivi - diminuisce il gettito. Quindi, se vi fosse stata una sorta di *fiscal compliance* (o strizza fiscale), quel gettito sarebbe dovuto in qualche modo aumentare. Certo che è aumentato il gettito IRES, cioè il gettito dell'imposta sulle persone giuridiche, ma perché? Perché è variata la normativa. Infatti, se si deve considerare come un reddito ciò che era un costo, un ammortamento o una spesa di investimento, è chiaro che la base imponibile aumenta molto, quindi aumentano molto anche le tasse che si pagano. Non a caso, i dati poi non quadrano con il gettito dell'IVA: questa aumenta in costanza di diminuzione, invece, del gettito dell'IRE. Il risultato complessivo è che, se vi fosse stato un adeguamento spontaneo dei contribuenti, avremmo dovuto vedere un aumento anche dell'imposta personale delle persone fisiche, cosa che non è accaduta. Ciò significa che la variazione nelle entrate non deriva da altro che, in primo luogo, dalla modificazione della base imponibile, che viene dal passato, dalla variazione della normativa in tema di fiscalità aziendale e, in terzo luogo - e lo vediamo con il dato IVA - dall'andamento spontaneo dell'economia, quindi la crescita che abbiamo avuto nel corso dell'ultimo anno. Crescita, però, che - come dicevo - difficilmente si potrà mantenere potrà mantenere anche nel futuro. Quindi, la *fiscal compliance* non esiste. Abbiamo avuto una situazione di miglioramento che deriva principalmente dal miglior andamento dell'economia, ma attenzione, perché la stiamo bruciando. Ulteriore dimostrazione del - se posso permettermi di definirlo così - di gestire l'assestamento è, sempre nell'emendamento del Governo, la voce che vede una diminuzione

nascondere la spazzatura sotto il tappeto e rinviare questo tipo di spesa al futuro, esattamente come sta facendo, ad esempio, con i contratti del pubblico impiego? Allora, cosa viene fuori? Un'operazione di *window* *dressing*, dalla quale le spese del 2007 in qualche modo risultano inferiori rispetto a quello che sarebbero effettivamente. Bastano solo due esempi: risorse proprie dell'Unione Europea, meno un miliardo e 300 milioni di euro, e rinnovo dei contratti del pubblico impiego, che viene fatto slittare all'anno prossimo.

che non possiamo condividere una simile impostazione dell'assestamento che non fa altro che mantenere un quadro nel quale si utilizza la leva delle entrate per alimentare la spesa, il che va in senso assolutamente contrario rispetto a ciò che dovrebbe fare

attuale tra far scendere prima le entrate o la spesa, credo che la tecnica americana di affamare la bestia sia forse quella migliore: prima bisogna far scendere le entrate e conseguentemente diminuire la spesa, altrimenti non riusciremo mai ad ottenere un risultato ragionevole, perché ci sarà sempre qualche motivo e qualche *lobby* che spingerà ad aumentare la spesa. Lo abbiamo visto per quanto concerne gli enti locali, dove con la finanziaria sono diminuiti i trasferimenti, ma sono aumentate le tasse e le addizionali locali che sono sempre pagate dagli stessi contribuenti italiani. Credo che lo vedremo anche con l'esplosione futura, checché ne dica il Governo che sostiene che nel 2007 si verificherà un risparmio: in realtà, credo che anche lì ci sia molta spazzatura sotto il tappeto. Per quanto concerne la spesa sanitaria è il momento, credo, di invertire la tendenza. Ma sarà difficile che questo Governo la possa invertire: dovremo aspettare il prossimo e spero che arriverà presto.

Presidente, i colleghi Ripamonti, Polledri e Baldassarri hanno fatto riferimento, nei loro interventi, all'assestamento: quindi, non spetta a me replicare. Per quanto attiene, invece, le considerazioni svolte dai colleghi Eufemi e Vegas, relative al rendiconto,

evitando di apprezzare anche gli elementi positivi, ma non mi pare che abbiano aggiunto nulla di nuovo rispetto a quanto contenuto nella relazione. Pertanto, credo che non ci sia alcuna ragione per svolgere ulteriori considerazioni in sede di replica.

svolgere alcune brevi considerazioni, anche per consentire la prosecuzione dei lavori. Mi sembra comunque opportuno fornire alcuni chiarimenti a quesiti che sono stati chiesti anche dai relatori. Per quanto attiene al rendiconto non c'è molto da dire, se non che si tratta di un esercizio di transizione. È stata avviata la riqualificazione della spesa in favore degli investimenti; è stata avviata un'azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale che già nel 2006 ha prodotto

trasparente e costituirà una indispensabile premessa per avviare una riflessione critica, congiuntamente con il Parlamento, sia sulle dotazioni finanziarie dei singoli programmi di intervento pubblico, sia sull'organizzazione amministrativa. Quindi, in questo posso assicurare che ci saranno sostanziali progressi. Per quanto riguarda alcuni puntuali chiarimenti chiesti in particolare dai relatori, in merito all'andamento dell'IRE e alle ritenute sul lavoro dipendente, la revisione al ribasso fondamentalmente rispecchia una revisione degli scenari e delle previsioni macroeconomiche. A giugno lo scenario prevedeva una crescita delle retribuzioni pubbliche dell'1,8 per cento e di quelle private del 6,8 per cento; alla luce degli andamenti effettivi degli incassi dei primi otto mesi, le retribuzioni dei dipendenti pubblici stanno segnando una flessione pari all'8,5 per cento - questo anche a dimostrazione dell'azione di contenimento avviata

esiste una componente flessibile, variabile di anno in anno, per cui, mentre vi è certezza sui minori contributi per quest'anno, non si può allo stato attuale dare con certezza che questa riduzione possa essere considerata permanente. Infine, l'aspetto forse più importante riguarda il nesso tra assestamento e obiettivi di politica economica e finanziaria. È opportuno ricordare come l'assestamento consenta di adeguare la rappresentazione dei fatti senza però che ci sia alcun nesso meccanico con gli obiettivi di politica economica. Nel caso in cui l'Esecutivo intendesse modificare gli obiettivi di finanza pubblica, la modifica verrebbe proposta al Parlamento con la Nota di variazioni al Documento di programmazione economico-finanziaria. Non ritengo quindi opportuno affrontare ora le questioni attinenti alla politica economica dell'anno 2008 e degli anni successivi, pur confermando i macro-obiettivi che caratterizzano la politica economica del Governo riassumibili nei tre obiettivi: risanamento, sviluppo ed equità.

desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo articolo 7, che rappresenta una vera e propria sanatoria rispetto alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultati in sede di consuntivo. Credo sia un atto piuttosto grave: è una violazione di legge, come ho già avuto modo di dire, alla quale la Corte dei conti si è ampiamente richiamata. Tale violazione merita di essere sottolineata e per questo annuncio il mio voto contrario sull'articolo in

Signor Presidente, desidero illustrare sinteticamente i motivi che inducono il Governo a presentare un emendamento all'assestamento. Come ho avuto modo di illustrare nell'ampio dibattito che si è svolto ieri in Commissione bilancio, inizialmente, il disegno di legge di assestamento, presentato a giugno, apportava alcune correzioni alle entrate tributarie coerenti con quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Successivamente, con l'emendamento presentato qualche giorno fa, i dati sono stati rettificati per tener conto degli incassi effettivamente introitati nei primi otto mesi, quindi a tutto agosto. Ieri, nel momento in cui ho avuto modo di replicare agli interventi svolti in Commissione, avevo accennato al fatto che ieri stesso si era reso disponibile il dato relativo agli incassi del mese di settembre teniamo presente che per quel che attiene i versamenti per autoliquidazione sono mesi particolarmente rilevanti - e avevo altresì accennato al fatto che il dato di settembre confermava l'andamento particolarmente favorevole dei versamenti di autoliquidazione per l'IRES, l'IRES, l'imposta sul reddito delle società. Ora, al fine di assicurare la massima trasparenza ed il rispetto del Parlamento, si ritiene opportuno presentare un emendamento all'assestamento al fine di allineare gli incassi tributari con quanto sarà presentato e illustrato al momento della discussione della Relazione previsionale e programmatica. Pertanto, così come vi era stata simmetria al momento della presentazione del disegno di legge di assestamento tra le entrate tributarie di allora e il Documento di programmazione economico-finanziaria, si ritiene opportuno, appunto per garantire la massima trasparenza e quindi per rispondere ad alcune delle osservazioni svolte durante la discussione, assicurare un'assoluta coerenza tra quanto verrà iscritto tra le entrate tributarie nel documento di bilancio e quanto risulterà nel quadro economico e finanziario che verrà illustrato nella Relazione previsionale e programmatica, che sarà presentata

grave per alcuni motivi che non sto qui a ricordare. Certamente è grave che l'emendamento sia stato presentato in Aula dopo l'approvazione del rendiconto e dopo l'esame in Commissione bilancio;

infrannuale prima della legge finanziaria. Per queste ragioni, credo, Presidente, che l'emendamento debba essere riportato all'esame della Commissione bilancio. Senatore Ferrara, la richiesta del Governo, a termini di Regolamento, non ha alcun significato se l'emendamento non c'è e quindi sembra più una richiesta di sospensione per produrre un effetto-annuncio, visto il vertice di maggioranza. Io inviterei quindi la Presidenza a non sospendere i lavori, a meno che il Governo non faccia un'esplicita richiesta di sospensione ai sensi del Regolamento, magari senza dire i motivi, ma non certo preannunciando la presentazione di un emendamento che non ha nessun significato al momento attuale.

Allo stato attuale, l'emendamento non c'è e pertanto la Presidenza non può neppure giudicare rispetto alla sua ammissibilità. Rispetto al fatto che arrivi, io credo che sia certo e quindi, alla luce di questo, il senatore Morando ritiene che nel momento in cui dovesse pervenire sia utile un esame da parte della sua Commissione? Presidente, devo confessare che non capisco perché dovrei intervenire in questo momento. Per quanto riguarda la Commissione bilancio, abbiamo esaminato tutti gli emendamenti presentati, li abbiamo regolarmente votati e siamo venuti in Aula con i relatori, come lei ha potuto constatare, assieme agli altri colleghi. Ho ascoltato anch'io l'annuncio che ha fatto il Governo, ma lei, ovviamente, non è in grado adesso di conferirmi, per esaminarlo in Commissione, un emendamento che non è stato presentato. Quindi, quella del Governo, che io interpreto come una proposta di sospensione dei nostri lavori per valutare la possibilità di presentare un emendamento, è una proposta che, come tale, dovrebbe essere valutata dell'Aula del Senato per quello che è. La Commissione bilancio per ora non deve fare nulla perché non c'è nessun emendamento presentato; quando sarà presentato, naturalmente, se l'emendamento ci sarà conferito per un parere, come assolutamente io devo

sono stati analizzati ieri ed io ho preso un impegno con gli uffici della Ragioneria generale dello Stato di poter presentare l'emendamento entro il termine dei lavori odierni, che era programmato per le ore 19 di stasera. Ora intendo anche verificare

Se ho ben capito, il Governo ha risposto alla sua domanda, dicendo che ritiene di poter presentare l'emendamento entro il termine di chiusura della seduta, che è fissato appunto alle ore 19.

la Presidenza è in grado di stabilire il termine per i subemendamenti e può chiedere alla Commissione bilancio di pronunciarsi anche in serata, in maniera che domani mattina

devo dire che provo comprensione nei suoi confronti, ma anche verso i colleghi della maggioranza, perché l'atteggiamento del Governo è veramente inqualificabile: che all'ultimo momento un rappresentante del Governo si alzi e dichiari che c'è l'intenzione di presentare un emendamento, francamente è la prima volta che nelle Aule parlamentari mi trovo ad ascoltare una dichiarazione del Governo di questa natura. Siccome ho comprensione, il Gruppo il Gruppo di Alleanza nazionale si rimette alla sua saggezza per cercare di sbrogliare questa matassa, creata esclusivamente dal rappresentante del Governo.

stante l'atteggiamento del Governo stesso. ha più volte richiamato nella seduta antimeridiana la Presidenza affinché il Regolamento in quest'Aula sia rispettato. Vorrei ricordare al senatore Boccia, al Governo, che è meno esperto del senatore Boccia, e a tutti i colleghi che la sospensione di una seduta

una richiesta di sospensiva. Questo è l'unico modo per sospendere la seduta. In caso diverso, signor Presidente, dobbiamo procedere alla discussione del disegno di legge di assestamento, così come è stato presentato. Non credo che, a termini di Regolamento, vi siano altre soluzioni.

la prego, vorrei rivolgermi non solo alla sua attenzione e alla sua intelligenza, ma anche al suo buon cuore. Cerchi di capire che siamo tutti impegnati ad approvare una manovra di assestamento di bilancio che - come le hanno spiegato prima gli autorevoli colleghi Baldassarri e Vegas - è difficile da approvare senza rendersi conto dell'evidente trucco dei conti. Il fatto che, nonostante questo si arrivi, a pochi minuti dal voto e dalla presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo, che lei ha già avuto modo di illustrare questa mattina in Commissione bilancio, all'annuncio che evidentemente i rapporti tra questo Governo e la Ragioneria generale dello Stato non sono poi così buoni. Forse perché persino alla Ragioneria generale dello Stato il vostro trucco dei conti non torna: nemmeno lì. Allora, la pregherei, sottosegretario Sartor, lei è di Verona, come sono di Verona io (è di Verona anche la nuova miss Italia, appena eletta): non ci faccia fare brutta figura. Grazie Sottosegretario, procediamo con i lavori se possibile. Presidente, la questione che ci viene sottoposta è di particolare delicatezza:

che, fatte salve le procedure di presentazione dell'emendamento, qualora fosse presentato, noi chiediamo alla Presidenza di rimettere il provvedimento in Commissione, per consentire alla Commissione il suo *iter* normale. È evidente che è proprio su quell'emendamento che si concentra l'intero dibattito e la discussione politica anche in Commissione. Pertanto, la richiesta che formulo è che, ove fosse presentato, il provvedimento di assestamento sia rimesso in Commissione per il suo normale *iter*. In via subordinata, se si può dire così, chiedo che la rimessione dell'emendamento in Commissione

francamente non comprendo le rimostranze dei colleghi dell'opposizione. Il sottosegretario Sartor ieri, in Commissione, ha preannunciato quanto ha oggi affermato in Aula, e cioè che il Dipartimento per le politiche fiscali (non la Ragioneria generale dello Stato) stava completando, nella giornata di ieri, il rilevamento delle entrate del mese di settembre e che quindi, con ogni probabilità, relativamente all'IRES ci sarebbe stata un'ulteriore maggiore entrata. Cos'altro avrebbe potuto fare il Governo se non presentare oggi (cioè un giorno dopo) un nuovo emendamento per aggiornare il dato contenuto in quello presentato alcuni giorni fa? Oppure avrebbe dovuto tacere questo dato?

Non credo ci si debba nascondere dietro un dito, è stata chiesta questa sospensione, l'argomento domani mattina lo riprenderò (se non viene il Presidente sarò ancora io a presiedere) e garantisco a tutti, con assoluta imparzialità,

Avverto gli onorevoli colleghi che, come comunicato per le vie brevi ai Gruppi, a conclusione della seduta antimeridiana di domani, si svolgerà un'informativa del Governo sulla situazione in Myanmar.

Come lei saprà e come avrà appreso anche dalle agenzie di stampa e dai giornali, il collegamento tra Lione e Torino non sarà realizzato perché, contrariamente a quanto detto in tutte le sedi

perché, se così è - e mi piacerebbe essere smentito - l'Italia verrà tagliata fuori dallo sviluppo delle comunicazioni europee e credo che gli italiani debbano saperlo. Quindi, il Governo deve rispondere.

Grazie,